Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca*: «Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5, recante disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011»

è certamente di grande importanza il fatto che il Parlamento intenda ancora una volta ascoltare il Governo su una situazione diversa da quella di cui parlammo la scorsa settimana, ma certamente ancor più drammatica e potenzialmente destabilizzante per l'intero bacino mediterraneo. la questione libica non è per la prima volta all'attenzione del Governo italiano e del Parlamento italiano. Il Governo Il Governo dell'Italia, non da oggi, ma almeno dall'inizio degli anni Novanta, cominciò a lavorare per la progressiva normalizzazione di un rapporto che aveva caratterizzato nei decenni la relazione italo-libica, con momenti di speciale difficoltà, con momenti talvolta di grave crisi, con momenti di vera e propria inimicizia e ostilità. Governi di diverso colore politico, con Primi Ministri anch'essi di diverso colore politico - e altrettanto per i Ministri degli affari

tutti quei Governo lavorarono - e abbiamo lavorato anche noi in questa legislatura - per definire un quadro che sostituisse l'inimicizia e il retaggio del colonialismo italiano sulla Libia con una nuova prospettiva di stabilità. Il Parlamento italiano condivise questa impostazione approvando il Trattato bilaterale con la Libia nel 2009, alla Camera con ampia maggioranza e in questa Aula del Senato, nel febbraio 2009, con la larga maggioranza di 232 voti a favore e di 22 voti contrari. È evidente che - come fu segnalato da coloro che intervennero nel Parlamento - era il segno della volontà dell'Italia nel suo complesso

mediterranea, migratoria e umana. Ricordate il grande problema dei profughi e degli esiliati (che, tra l'altro, nell'ambito di questo accordo ancora non ha trovato, a mio personale avviso, la completa soddisfazione). Allora è evidente che se questo accadde, accadde perché anche in Europa qualcosa era cambiato, anche in Europa ci si era resi conto che la Libia, Paese mediterraneo, doveva essere ricondotto ad un quadro negoziale con l'Unione europea. Quando giustamente, sulle colonne di un grande giornale, qualche giorno fa il presidente Prodi rivendica il merito di aver sdoganato in Europa la Libia, lo fa riconoscendo che in quel momento storico la strada che i Governi stavano percorrendo era quella giusta. Oggi la situazione è completamente cambiata. Abbiamo di fronte a noi una situazione drammatica, anzi estremamente drammatica, in cui il bagno di sangue annunciato ieri da Gheddafi segue le morti già viste, testimoniate, constatate nelle strade, non soltanto della provincia della Cirenaica, ma anche di Tripoli, con *raid*, uccisioni, mitragliatori in azione nelle strade, e con un numero di morti che ancora non siamo in grado di quantificare. Fonti non confermate hanno parlato di 1000 morti; altre fonti hanno dato indicazioni superiori.

È evidente, quindi, che la situazione libica, con una regione, quella della Cirenaica, ormai fuori dal controllo delle autorità di Tripoli e con altre regioni (la Tripolitania, in particolare, dove scontri violenti ci sono stati e saranno certamente in corso presto), ci mostra l'immagine di un Paese in uno stato di guerra civile, con le autorità della capitale che ordinano attacchi contro lo stesso popolo libico, bombardamenti e azioni di violenza inaudita. È evidente che questo potrà avere e avrà un impatto - come detto - destabilizzante, non solamente per le relazioni con l'Italia. Avete ascoltato ieri persino parole che hanno riecheggiato la retorica anti-italiana e anti-americana, un discorso televisivo in cui da Tripoli Gheddafi ha accusato l'Italia e gli Stati Uniti di essere fomentatori delle sommosse, e addirittura l'Italia di avere fornito razzi ai rivoltosi: notizia, come è ovvio, assolutamente falsa, ma che dà l'idea di un degradarsi della situazione e anche dei rapporti. Questo - ed è la prima riflessione che desidero fare - per l'Italia pone immediatamente l'esigenza di una riflessione politica. Dovremo affrontare nelle prossime settimane una questione complessa, che credo sarà drammatica non solo per l'Italia, ma per l'intera Europa. Essa riguarderà certamente anzitutto la dimensione umana, di di cui parlerò, quella migratoria in particolare; la dimensione della collaborazione economica, che riguarda migliaia e migliaia di famiglie italiane dipendenti da aziende, imprese che hanno investito, investiranno nelle loro previsioni e forse non potranno più investire nei rapporti economici con la Libia; la questione energetica, della quale pure dirò. Il tutto richiederà una seria valutazione dell'interesse nazionale italiano a dare una risposta a questa drammatica crisi in cui ci stiamo incamminando e di farlo - a mio avviso - nell'unità del Paese. Questo è il primo punto che intendo toccare. Sono certo che, come si fa e si deve fare nelle grandi democrazie quando una questione tocca la politica estera, e, ancor più profondamente, l'interesse nazionale del Paese, la maggioranza e tutte le forze di opposizione che si rendono disponibili dovranno e potranno insieme raccogliere informazioni, consultarsi reciprocamente, lavorare insieme per definire momento per momento quale sia il modo migliore per tutelare l'interesse nazionale: non l'interesse del Governo italiano in carica. L'interesse nazionale, a mio avviso, si ricerca anzitutto attraverso un lavoro forte con il Parlamento. Non posso evidentemente dire a voi quale ne sia la modalità: il Presidente del Senato (e lo stesso ho detto oggi al Presidente della Camera) e voi parlamentari valuterete le forme,

di riunire in permanenza l'Ufficio di Presidenza per una consultazione ed uno scambio di informazioni costante con il Governo, il Governo non solo non si sottrarrebbe Questo potrebbe comportare il coinvolgimento di organi parlamentari istituzionali, alcuni dei quali presieduti da esponenti dell'opposizione. Onorevoli Onorevoli senatori, questo è l'avviso del Governo relativamente ad una prospettazione politica

che non può dividerci, ha formulato un appello a lavorare insieme. Questo appello il Governo lo raccoglie con convinzione, perché credo che si debba mettere da parte l'occasione e l'opportunità - che qualcuno può avere considerato e può considerare - di usare questioni di politica estera così delicate per ragioni di lotta politica interna. Qui l'interesse nazionale prevalente è lavorare insieme per definire le prossime mosse, di cui poi credo tutti noi dovremo rispondere ai cittadini italiani e di cui il Governo - questo sì - ha la responsabilità di rispondere dinanzi alle istituzioni internazionali. internazionali. Onorevoli senatori, la situazione - come accennavo - è stata rappresentata pubblicamente e in colloqui e contatti che abbiamo avuto in molti modi.

aveva telefonato per aggiungere la sua voce a quella del segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon. Il leader di Tripoli ha parlato in questi giorni con il presidente Berlusconi e con il Segretario generale dell'ONU, e ad entrambi, che gli chiedevano ovviamente la condanna e la cessazione immediata delle violenze sul popolo libico, ha risposto facendo riferimento a quello che poi ha affermato: l'azione di gruppi isolati, il pericolo del fondamentalismo islamico nella Libia orientale e la volontà di andare avanti. Onorevoli senatori, a tutto c'è un limite.

può essere mai in alcun modo giustificata: nessuna spiegazione, nessuna motivazione, nessuna scusa. Lo abbiamo chiesto e lo ripetiamo nelle sedi internazionali, unendoci e rappresentando con l'Unione europea una voce chiara e unanime: condanna senza riserve di queste azioni, richiesta immediata di sospensione delle violenze per aprire un dialogo nazionale e per ascoltare la voce del popolo. Questa è stata la reazione dell'Europa, questa è stata la reazione dei nostri amici americani, questa è stata in Italia la forte volontà che il messaggio del Capo dello Stato ha voluto trasmettere con la sua pubblica dichiarazione, e la voce che il Governo ha evidentemente rappresentato e rappresenterà. Ieri, al Cairo, incontrando il Segretario generale della Lega araba, ho avuto la possibilità di avere da lui in anteprima il testo che sarebbe poi diventato la dichiarazione di condanna della Lega araba per i comportamenti posti in atto dalla *leadership* di Tripoli: una condanna ferma, unanime di tutti i Paesi della Lega araba, che hanno voluto dal mondo arabo fare unire la loro voce alla voce di condanna per le violenze, gli spargimenti di sangue, il rischio di guerra civile, il rischio - in altri termini che quel Paese si trasformi davvero in un luogo dove avvengono stragi, dove il popolo si divide e dove la guerra civile purtroppo viene alimentata, fomentata, incoraggiata. La Lega araba ha detto una parola importante a cui stanotte si è aggiunto, da ultimo, il Consiglio di sicurezza dell'ONU. Il quadro internazionale ormai è chiaro, credo che da questo quadro internazionale dobbiamo partire, dandolo ormai come la posizione consolidata cui tutti i Paesi del mondo - come detto si atterranno. Oggi non voglio ricordare appelli a cessare la violenza, che sono provenuti persino da Paesi in cui purtroppo le violenze si stanno verificando e si verificano con estrema gravità e che pure hanno trasmesso questo messaggio. Ma, insomma, se l'Unione europea, gli Stati Uniti, la Lega araba, il Consiglio di sicurezza dell'ONU questo hanno detto, credo che mai nella storia della politica estera recente vi sia stata una tale comunanza di intenti nella comunità internazionale. Qual è la situazione che abbiamo davanti? Abbiamo davanti un'opposizione libica magmatica. La storia della Libia, per chi la conosce, insegna di divisioni storiche tra gruppi tribali. Alcuni di questi gruppi tribali hanno già agito contro il regime di Tripoli, hanno già dichiarato di voler sostenere le azioni di coloro che sono nelle strade, che chiedono libertà, che chiedono diritti, che chiedono un cambiamento. Non abbiamo visto ancora emergere, come è pure emersa in alcuni dei Paesi attraversati dal vento di libertà nel Mediterraneo del Sud, una *leadership* coesa dell'opposizione. È un elemento su cui dobbiamo riflettere, considerando che nella Cirenaica esistono gruppi che sono certamente ispirati da motivazioni radicali islamiste, anche se sarebbe sbagliato dire che l'azione contro il Governo di Tripoli è nata con motivazioni radicali islamiste: è nata dalla volontà, dalla richiesta forte, non di pane perché la Libia non è un Paese povero, ma di diritti, di libertà, di cambiamento. La seconda riflessione importante che desidero fare con voi è la significativa moltiplicazione delle defezioni da un Governo che appariva solo fino a qualche giorno fa straordinariamente unito e coeso al suo interno, tanto da sollecitare e da rappresentare alla stessa Unione europea fino a 20 giorni fa la volontà di definire molto presto il negoziato per un accordo quadro tra Libia ed Unione europea. Ebbene, abbiamo visto le dimissioni del Ministro della giustizia, del Ministro della sicurezza di Bengasi (che si troverebbe ora a Bengasi); abbiamo visto la defezione del Vice capo delle Forze armate libiche, di molti diplomatici in giro per il mondo. Le Forze armate in Libia non hanno la struttura delle Forze armate egiziane;

di alcuni squadroni, di alcuni piloti, di alcuni equipaggi di navi, che hanno dichiarato di ribellarsi agli ordini di sparare contro il loro stesso popolo. Si tratta di una situazione magmatica.

piuttosto significativa, a quelle che invece riportano immagini di sparatorie, echi di bombardamenti anche nei quartieri periferici della capitale. Credo che, dinanzi a questo, ancora una volta la reazione della comunità internazionale non si possa fermare. L'Italia sosterrà in un quadro europeo le ulteriori appropriate misure che verranno decise - non sappiamo ancora quali, ma le stiamo esaminando nel tavolo tecnico europeo - per fare fronte alla sconsiderata eventualità che la violenza non si fermi e che le morti di civili innocenti continuino.

È un dato di fatto che molti di voi conoscono. In Libia abitano circa 7 milioni di persone, di cui 2,5 milioni non sono cittadini libici, sono persone provenienti da altri Paesi, in particolare dell'Africa sub-sahariana, che risiedono in Libia perché hanno un lavoro, spesso misero, modestissimo, ma che consente loro di vivere in

continuazione della crisi, come una delle conseguenze più pericolose per l'equilibrio dello Stato egiziano in transizione: ricordo che la provincia occidentale egiziana è al confine con la provincia orientale della Libia, cioè la Cirenaica. L'Egitto è preoccupato,

di cercare fortuna imbarcandosi verso Nord; se questa piccola percentuale fosse solo del 10 per cento, si tratterebbe di 250.000 potenziali immigranti verso le coste dell'Europa. Ciò

di un coordinamento delle azioni e di una più forte azione per la prevenzione: è ora che l'Europa - questa sarà la voce che porterà domani il ministro Maroni a Bruxelles al Consiglio dei Ministri dell'interno e della giustizia - prenda il coordinamento e la gestione dell'eventuale impatto di un flusso migratorio che né l'Italia né

Anonimi funzionari di Bruxelles già ci fanno sapere che ci daranno 100 milioni di euro, che lavoreranno con la missione di pattugliamento Frontex, ma che gli immigrati che arrivano in Italia rimarranno in Italia, che quelli che arrivano a Malta rimarranno a Malta.

siete voi, vorrei più Europa non meno Europa. Credo che l'Europa debba dire, senza se e senza ma, che se si dice no all'Italia, a Malta e alla Grecia in questo momento si rompe il pilastro della solidarietà europea

fare. Credo che tutta l'Italia debba essere convinta che noi non parliamo altro che di un'Europa che faccia l'Europa, di un'Europa che si assuma la responsabilità, così come ha fatto per la protezione dei mercati e dell'euro e anche per la difesa delle banche. Vogliamo accettare l'idea che l'Europa non si preoccupi

sono rientrati, solo da Tripoli, 650 connazionali. Siamo in contatto con connazionali in alcune città,

stiamo organizzando il loro rientro in Italia, mentre 150 impiegati dell'ENI sono rientrati con voli dell'azienda. Abbiamo oggi una stima generale di un migliaio di italiani in tutto il territorio libico. Certamente la situazione più delicata è quella della regione orientale, la regione di Bengasi, dove il primo aeroporto è chiuso e il secondo, quello di Misurata, è egualmente nell'impossibilità di funzionare: lì abbiamo circa 180 italiani in attesa di partire. di partire. Una nave italiana, partita 27-28 ore fa, si appresta ad avvicinarsi ai porti della regione di Bengasi,

in contatto con le autorità della Difesa, con il COI, per la gestione di un volo C-130), con alcuni equipaggiamenti speciali e con alcune squadre di pronto intervento di sicurezza che, atterrando a Tripoli, potranno garantire,

sanitarie, quindi la Croce Rossa. Siamo pronti a promuovere un canale umanitario italiano verso la regione di Bengasi, dove i rapporti e le informazioni che cominciano ad arrivare con l'arrivo di giornalisti occidentali - lo avete letto anche sui giornali italiani - parlano di ospedali saturi, di necessità di sangue per le trasfusioni, di morti per le strade. Io credo che l'appello che ci è stato rivolto dalla organizzazione medica delle comunità arabe stamattina debba essere raccolto. Abbiamo avuto il primo, importante via libera: la Federazione italiana dell'Ordine dei medici è pronta, con medici volontari. Ci stiamo lavorando. Mi auguro che riusciremo in brevissimo tempo, chiedendo chiedendo eventualmente lo sgombero dell'aeroporto e della pista di Misurata, ad attivare quel canale umanitario italiano con la Croce rossa, con i medici volontari, con i medici locali, che potrebbe portare almeno in quella provincia, che è stata così duramente ed orribilmente colpita, qualche aiuto medico di primissima necessità. Vi è un impatto sulla situazione energetica. Non mi dilungo molto perché il ministro Romani è stato oggi anche pubblicamente molto chiaro: la fornitura di gas libico sospesa è stata già rimpiazzata per le esigenze ordinarie da un aumento di fornitura, avendo l'Italia una buona diversificazione di approvvigionamenti, dall'Algeria fino alla Russia. Quindi, questa situazione non avrà un impatto negativo sul fabbisogno energetico italiano. Certamente vi sarà un impatto sul settore industriale infrastrutturale. L'insieme dei contratti che imprese italiane, con i relativi dipendenti, avevano già negoziato supera i 4 miliardi di euro. evidentemente che soffrirà, se non si ripristineranno in tempi rapidi condizioni accettabili per il lavoro e per la operatività dei cantieri nelle imprese italiane. È un altro degli aspetti di cui il sistema Italia dovrà discutere insieme, ovviamente con la comunità imprenditoriale. Concludo il mio intervento dicendo che le richieste puntuali che noi abbiamo già fatto all'Europa non si limitano a questo, non si limitano a questo, ma si estendono alla proposta operativa che l'Europa, attraverso Frontex, l'agenzia europea, assuma il vero e proprio controllo di gestione dell'andamento dei flussi, anche sulla base di direttive europee, che sono del 2008, ma sono entrate recentemente in vigore in tutti Paesi europei. Sono direttive - qualcuno dei colleghi della Camera ha oggi notato - non ancora ratificate dall'Italia. Non vorrei fare offesa alla cultura giuridica del Senato se ricordo che queste direttive sono immediatamente operative perché sono puntuali. Con il nuovo ordinamento, dopo il Trattato di Lisbona, si tratta di direttive che, anche se non formalmente ratificate nei loro principi, sono immediatamente applicabili, e certamente sono applicabili a Frontex, l'agenzia europea, che per prima ha il dovere di rispettare una direttiva recentemente entrata in vigore. Questo è il quadro nel quale io chiedo al Senato di condividere, se lo vorrà, l'appello ad un lavoro comune Parlamento-Governo per l'informazione e la consultazione su questo grande tema che riguarda l'interesse nazionale dell'Italia, dicendo con assoluta certezza che si è superato ogni limite sulla accettabilità e sulla giustificabilità di comportamenti che stanno offendendo in queste ore i diritti umani basilari, e che niente mai potrà giustificare o perdonare. *(Applausi

dal punto di vista della politica internazionale, di fronte ai tanti che leggiamo in questi giorni sui giornali e di fronte ai molti che ascolteremo in questo dibattito. Tuttavia, volevo in qualche modo sottoporvi la riflessione di un senatore di fila (di ultima fila, se mi è concessso dirlo), di un cittadino qualsiasi, che è stato chiamato per qualche anno a dare il proprio contributo alla legislazione e alla politica di questo Paese e al quale in questi anni è stato richiesto di accettare, quasi di ingoiare, per superiori ragioni di Stato, non solo le comprensibili esigenze imposte geograficamente da un vicino scomodo, ma

anche in questa città: le tende nei giardini romani, il baciamano reso dal Presidente del Consiglio (al quale anche i suoi detrattori non vogliono così male da considerarlo alla stregua del dittatore libico), il codazzo delle amazzoni e la lezione sull'Islam resa alle giovani adepte italiane. Io sono felice che il Senato, a suo tempo, sia riuscito a negare quest'Aula per uno *show* di Gheddafi, che si è poi svolto in un'altra sala del Senato sala, dopo un'attesa assai lunga, i senatori sono stati costretti ad ascoltare gli sproloqui vagamente ricattatori di un dittatore autoritario che oggi, in spregio a qualunque regola di democrazia, rifiuta l'evidente volontà del suo popolo di scegliersi un'altra guida e impone, con la sua volontà di potere, il sacrificio e il sangue a migliaia di suoi compatrioti. compatrioti. Io mi chiedo se fosse necessario questo: se gli evidenti e importanti interessi dell'Italia e dell'Europa, la presenza di molte nostre aziende e di molti nostri connazionali, la strategicità dei rifornimenti energetici richiedessero tutto questo. Io do atto al Presidente del Consiglio di avere finalmente e chiaramente preso le distanze,

mosso certe critiche per tempo, tuttavia vorrei che oggi la situazione che si è creata non rappresentasse lo strumento e il pretesto per una strumentalizzazione politica ad uso interno. Di questo non c'è bisogno, quanto, forse, potrebbe anche essere stato perseguito con metodi sbagliati era, ed è, l'interesse dell'Italia, dell'Europa e dell'Occidente. Di fronte a questo interesse, ciò che dobbiamo fare noi oggi noi oggi è contribuire ad assicurare una transizione democratica del regime libico verso un assetto che non faccia prevalere altre istanze non democratiche, legate, per esempio, al fondamentalismo religioso, e che, invece, consenta di superare questo difficile momento.

Signora Presidente, purtroppo dalle parole del Ministro non è arrivata un'oncia, che fosse una, di autocritica. Sicuramente si è molto parlato di interesse nazionale, ma occorre ricordare che l'Italia, l'Europa e l'Occidente si fondano sul diritto internazionale. Noi abbiamo degli obblighi precisi che derivano non soltanto dalla nostra Costituzione, ma anche dalle organizzazioni regionali e internazionali di cui facciamo parte: sicuramente l'Unione europea e altrettanto sicuramente l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Occorre quindi inquadrare in questo contesto, quello dello Stato di diritto a livello internazionale, ciò che avviene in questi giorni e rifarsi ai principi. principi. Pertanto, a livello nazionale occorre immediatamente sospendere questo maledetto e infame Accordo Italia-Libia per togliere la legittimità a quel signore; un signore che in questo momento in cui parliamo sta ammazzando i propri concittadini. Il Ministro ha parlato dello sforzo europeo necessario per accogliere i migranti o le persone che fuggono. Ebbene, anche in questo caso l'Italia, in virtù della vicinanza e della responsabilità politica che porta che porta nei confronti della Libia e degli altri Paesi nordafricani, deve giocare un ruolo fondamentale, anche perché a suo tempo, quando ci fu lo stesso tipo di problemi nella ex Jugoslavia, l'Italia non si candidò, come la Germania, ad ospitare oltre mezzo milione di jugoslavi a casa propria.

che ha anche annacquato la posizione comune dell'Unione europea, deve invece recuperare non solo parte del coraggio, che però mi pare non sia purtroppo tornato ad albergare nel nostro Governo, ma anche l'attenzione che da sempre ha nel rispetto e nella promozione dei diritti umani e fare almeno due cose: da una parte, imporre, assieme a tutto il resto della comunità internazionale, una *no fly zone* sopra la Libia, perché è proprio dall'aria che vengono ammazzati i libici; dall'altra, insistere perché si possa portare avanti una commissione d'inchiesta internazionale. internazionale. Signor Ministro, lei ci ha ripetuto più volte che nel 2005 è stato codificato il cosiddetto principio della responsabilità a proteggere. In virtù di quel principio, che deriva dai capitoli VI e VII della Carta delle Nazioni Unite le sue fondamentali articolazioni, noi dobbiamo intervenire per porre fine

che siamo il Paese più esposto in assoluto nei confronti della Libia, abbiamo fino ad ora intrapreso la politica giusta? Mi permetto

già da prima. So bene che ora noi descriviamo le cose fatte: ma noi abbiamo fatto la politica giusta? È stata giusta la politica che abbiamo fatto finora,

le prime avvisaglie? L'abbiamo capito noi che siamo normali parlamentari e l'abbiamo riportato in Commissione davanti a persone autorevoli.

*(IdV)*. Signora Presidente, ho ascoltato con attenzione le parole del Ministro e, come sempre, mi aspettavo qualche cosa di più incisivo e una reazione forse più coraggiosa. A pochi giorni dall'ultima

continua a non avverarsi. Come Italia dei Valori, pertanto, avremmo voluto che in Aula ci fosse stato oggi il presidente del Consiglio Berlusconi, e non il ministro Frattini, a riferire sulla posizione italiana sul genocidio che si sta compiendo in Libia. Infatti, non è stata la diplomazia della Farnesina, ma il *Premier* in prima persona a determinare la politica estera di totale asservimento dell'Italia a Gheddafi e - quindi - la nostra indiretta complicità con il bagno di sangue in atto a Tripoli. È al Presidente del Consiglio (quello che non c'è, quello che si è presentato in Aula solo tre volte dall'inizio del suo Governo, e soltanto per incassare qualche voto di scambio per ottenere una fiducia) che chiediamo delle spiegazioni. È sempre a lui che chiediamo la fine dei rapporti di sudditanza o di complicità con questo assassino, il *rais* Gheddafi. Dopo la compromissione dell'Italia con una dittatura a cui abbiamo dato 5 miliardi a cui abbiamo delegato la nostra politica sull'immigrazione e a cui abbiamo permesso di acquisire quote rilevanti delle maggiori imprese italiane - da Unicredit, a Finmeccanica e Capitalia è Berlusconi che deve assumersi la responsabilità di intervenire personalmente in Aula per fare direttamente, e non per procura, il *mea culpa* sulle relazioni pericolose intrattenute fino a poco fa con Gheddafi. che nella mia replica mi rivolgerò al presidente Berlusconi e non all'emissario ministeriale inviato in quest'Aula, che non rappresenta nulla più del portantino: così è stato definito dalla diplomazia americana nei tabulati di Wikileaks. Cari colleghi, sul bagno di sangue in Libia, sul genocidio di mille e più persone e sulla persistente violazione dei diritti umani, abbiamo sentito dal nostro Governo, non una condanna netta,

Il 23 dicembre scorso Berlusconi ha affermato: «Sono legato da amicizia vera con il presidente egiziano Mubarak, con il presidente libico Gheddafi e con il presidente della Tunisia Ben Ali». Di fronte al bagno di sangue che ha coperto l'intero Mediterraneo, oggi queste affermazioni varrebbero da sole le sue dimissioni, Presidente del Consiglio.

e il contrasto all'immigrazione clandestina verso l'Italia offerto dalla Libia, fosse giusto rispettare la sovranità di Tripoli, anche quando la sovranità si trasforma in atrocità. Ecco il motivo per cui ci indigniamo. Noi

Noi non vogliamo criticare anche una parte politica che ha votato il trattato di amicizia; vogliamo solo

il Presidente del Consiglio ha tenuto con Gheddafi un profilo da imprenditore, e non da Capo di Stato. Ha parlato di calcio, automobili, banche e aerospazio, gli interessi principali di Gheddafi e suoi.

ma sicuramente l'Italia tutta festeggerà il ritorno alla libertà.

In sostanza, al di là della diversa e profonda differenza di valutazione sulla linea di politica estera tenuta dal vostro Governo nel rapporto con Gheddafi, che è cosa diversa dalla Libia, riteniamo che si sia in presenza di un'emergenza nazionale ed internazionale che impone un supplemento di responsabilità da parte di tutti, nonché l'esigenza di fare in modo che la politica, per quel poco che ancora risulta credibile ai cittadini, sia nelle condizioni di salvaguardare gli interessi economici profondi che questo Paese ha in Libia e in quell'area geografica tormentata e di recuperare forza ed autorevolezza per porre in sede europea il problema di questo difficile e, per così dire, controverso rapporto con la Libia, ma anche con tutto ciò che nel bacino del Mediterraneo si sta

il Gruppo IdV e la componente dei radicali, ci siamo opposti al Trattato di amicizia italo-libico; lo abbiamo fatto non per una posizione strumentale e non perché non riconoscessimo e non riconosciamo l'esigenza di un dialogo, che peraltro ha una sua continuità di politica estera, che attraversa Governi della prima e della seconda Repubblica, di centrodestra e di centrosinistra, riguardando però accordi di cooperazione, che erano e sono settoriali. Cito, ad esempio, il caso dell'accordo in merito al quale tanto si polemizzò anche in quel periodo, il cosiddetto accordo riservato Dini, che riguardava la cooperazione tra il nostro Paese e la Libia in materia di polizia di frontiera, di contrasto all'immigrazione clandestina e così via. Tutto questo non è in discussione; non lo è mai stato, dal nostro punto di vista, ma era chiaro che l'idea di costruire un rapporto istituzionale forte attraverso un trattato sottoscritto con un soggetto che, per sua stessa ammissione, nelle sue ultime farneticazioni, Stato non è - mi riferisco al leader Gheddafi avrebbe posto una serie di problemi e criticità, non solo dal punto di vista del rapporto e della necessaria collaborazione sul fronte del contrasto all'immigrazione clandestina.

e che oggi la Libia, per la condizione in cui si trova e in cui è sempre stata, cioè nell'assenza di una dimensione statuale, non può garantire e non ha garantito. Ricordo a me stesso che uno dei problemi riscontrati in rapporto con l'immigrazione clandestina che proviene da quel canale è quello dell'identificazione, poiché la Libia non dispone di uffici anagrafici tali da consentire il rimpatrio attraverso l'identificazione dell'immigrato che viene dalla Libia. C'è un problema enorme, e su questo tema in quel trattato, posto che un trattato determina in legame sotto il profilo dei due ordinamenti giuridici, avremmo dovuto chiedere di più e qualcosa di diverso. L'altra questione che abbiamo posto e che torna di attualità riguarda l'articolo 4 di quel Trattato, che ha ad oggetto l'obbligo della non ingerenza negli affari interni. Noi ci siamo impegnati, sempre nel rispetto della legalità internazionale,

forse anche *ultra petita*, una *leadership*, eccessiva nel rapporto con questo personaggio che carica di responsabilità noi, perché dobbiamo con forza e con tutta l'autorevolezza possibile e immaginabile, che può venire solo da un fronte unitario di questo Parlamento, porre agli altri leader europei il tema della questione libica e dell'immigrazione. Anche questo è collegato peraltro alla questione relativa alla sicurezza energetica italiana e alla sicurezza degli interessi economici che noi abbiamo, forti e importanti, Per queste ragioni, signor Ministro, riconfermiamo le cose che abbiamo già detto e riteniamo che sia opportuno che il Governo e il Presidente del Consiglio si assumano la responsabilità, un po' meno coreografica e un po' più concreta, d'investire direttamente e con la propria persona, avendo un mandato da tutti i noi, di tutto il Parlamento, l'Europa della responsabilità di un intervento chiaro e netto su queste vicende, con un solo presupposto: la condanna senza se e senza ma di tutte le violazioni dei diritti umani che in questi periodi sono stati compiuti in quel Paese e la necessità di far cessare con ogni mezzo tutto ciò che lì sta avvenendo, perché diventa un'ulteriore miscela esplosiva, che non serve né ai Paesi del Mediterraneo, né all'Italia, né all'Europa, né al mondo. Signora Presidente, signor Ministro, colleghi, ci sono stati nei decenni scorsi molti momenti alterni nelle relazioni tra

ad oggi, ad avere mosso un attacco convenzionale e militare nei confronti dell'Italia. Un attacco *sui generis,* certamente. Fu nell'aprile del 1986, quando furono lanciati due missili sull'isola di Lampedusa. Dal '45 ad oggi l'Italia non ha subito attacchi militari al proprio territorio e, ancorché quello fosse stato all'epoca anche minimizzato dal nostro Governo Gheddafi chiarì che non aveva inteso colpire il territorio italiano, bensì una base americana che si trovava a Lampedusa - in quell'episodio, signor Ministro, io rintraccio tutte le contraddizioni, le criticità e le difficoltà dei nostri rapporti internazionali e dei rapporti bilaterali con la Libia. Questi rapporti sono fatti di due grandi filoni: il primo, che potremmo chiamare della necessaria razionalità, sia pur di fronte ad un interlocutore un interlocutore irrazionale e bugiardo, visto che lei stesso così ha definito Gheddafi nell'Aula della Camera dei deputati, signor Ministro, poco fa a proposito delle dichiarazioni da egli rese concitatamente nella giornata di ieri, in cui accusa l'Italia di avere armato i rivoltosi, oltre a sostenere che: «Ci siamo fatti rispettare da tutti: quando sono andato in Italia hanno salutato con rispetto Gheddafi», poiché «anche l'Italia è stata sconfitta dalla Libia». Questo è quanto ha dichiarato ieri il leader della rivoluzione libica. Ora, della parte necessaria e razionale, signor Presidente, signor Ministro, fanno parte le questioni che riguardano gli approvvigionamenti energetici, la sicurezza delle nostre frontiere, il controllo dell'immigrazione clandestina e, naturalmente, un contemperamento degli interessi economici nazionali anche con riferimento ad aziende che operano in Paesi a rischio, inclusa la Libia.

della Repubblica ha approvato una relazione, nell'aprile del 2009, nella quale si fa riferimento non soltanto a tutti i porti dai quali sono partiti, attraverso attività anche corruttive interne al regime libico, i clandestini, ma anche al giro di affari per ciascuno dei clandestini imbarcati all'epoca. Dunque, non vi è dubbio che da parte dell'attuale Governo la prosecuzione delle politiche, come il Ministro ha ricordato, intrattenute dall'Italia per cercare di limitare e di governare questo flusso ha avuto anche sostegni da parte dell'opposizione nella misura in cui si legava all'applicazione dell'intesa bilaterale che fu promossa dal ministro Amato, membro del Governo precedente, di questa attività, di questo sforzo e di questo tentativo - a nostro avviso - non ha fatto parte un'applicazione dei respingimenti che, in alcuni momenti topici, ha certamente violato accordi internazionali fondamentali in materia di diritti umani. Al contempo, tutti noi abbiamo dovuto agire, signora Presidente, perché queste politiche rispondessero a primari interessi della sicurezza nazionale. E' così per quanto riguarda la questione energetica e le aziende

che hanno oggi nei loro pacchetti azionari un'importante partecipazione libica, tale da assumere una dimensione strategica. C'è poi un lato irrazionale, signor Ministro, e di questo lato sono fatte alcune delle scelte a cui abbiamo assistito negli ultimi due anni. Penso che l'Italia abbia dei simboli nazionali, repubblicani, indisponibili e che il vostro Governo li abbia colpevolmente resi disponibili. Mandare le Frecce tricolori a Tripoli è stata una vergogna nazionale. Mandare le Frecce tricolori, e solo all'ultimo momento accettare autorevoli consigli che sconsigliavano che, anziché il fumo tricolore, esse producessero un fumo di colore verde intonato alla rivoluzione di Gheddafi è stata una pagina umiliante, come è stato umiliante destinare i corpi di *elite*

Allora, se questi sono i fatti, il lato della razionalità ci deve sempre guidare, ma l'insegnamento, signor Ministro, della dignità nazionale rispetto ai comportamenti

chiediamo formalmente al Governo di applicare le previsioni dello Statuto della Regione siciliana e di inserire la Regione stessa nell'unità di crisi, poiché quella terra è direttamente responsabilizzata nel quotidiano e nelle sua attività di Governo per quanto riguarda il flusso dei migranti. Dunque, il Governo deve compiere

Sappiamo che i nostri servizi informativi forse sono stati troppo *embedded* nel regime locale e non ci hanno consentito di ottenere informazioni tempestive e adeguate. Ecco perché, signora Presidente, signor Ministro,

cortocircuiti nelle relazioni con l'Europa. Apprezzo la dichiarazione del Ministro di voler cambiare rotta, ma su questi quattro punti (il coinvolgimento della Regione Siciliana, un impegno immediato per anticipare gli eventi, dato che - come il Ministro ha detto la volontà di dialogare con le forze in grado di costruire una equilibrio diverso nella Libia di domani e, infine, la possibilità di collaborare con l'Europa e la comunità internazionale) ci aspettiamo di più che non l'attendismo tenue che oggi ha esposto in modo, a mio avviso, inadeguato il ministro Frattini.

I problemi nascono proprio da ciò, perché una cosa è gestire i siti informatici, altra cosa è gestire masse in momenti estremamente delicati.

non hanno grossi supporti in periferia, mentre le città da sole non riescono a fare la differenza. Quello che ci tocca in questo momento da vicino è la Libia. Lì la situazione è molto diversa: la ribellione alla dittatura è stata molto estesa, e adesso anche le tribù delle zone interne e della montagna hanno aderito in massa alle proteste, e anche la Cirenaica, che non aveva mai visto di buon occhio

I militari - aspetto importante - hanno in parte disertato, disubbidito agli ordini. Gheddafi è ricorso in parte a mercenari, però, lì, ormai, l'epilogo sembra certo. Le accuse che sono state avanzate in quest'Aula non sono decorose, nel senso che le relazioni che ha intrattenuto l'Italia nei confronti della Libia e del dittatore sono state quelle obbligate nei confronti, ahimè, di chi governa uno Stato.

D'Alema, nonché a Prodi; D'Alema lo abbiamo visto addirittura abbracciare con disinvoltura terroristi di Hamas, con la giustificazione che in ogni caso bisogna tenere rapporti diplomatici.

Altro punto: distrattamente o meno, in un sistema di libero mercato ci troviamo grossi gruppi imprenditoriali italiani con importanti partecipazioni libiche. Iniziamo a pensare a questo. Un aspetto che non è stato rilevato e che, ad onor del vero, va messo sull'altro piatto della bilancia

della rivendicazione libica mai sedata contro il colonialismo italiano, che però con una cifra irrisoria spalmata su vent'anni, non in denaro ma in commesse italiane (pertanto, denaro che sarebbe ritornato ad imprese italiane) abbiamo tamponato una situazione, in cambio della quale abbiamo ottenuto la possibilità di perlustrare, con mezzi italiani, e, chiaramente, con personale militare misto le acque territoriali libiche, e abbiamo fermato quel flusso di immigrazione che dal Sudan, dal Ciad, dal Niger, dalle aree ad alta tensione umanitaria percorrevano la Libia, non per fermarsi in quel Paese ma per approdare in Europa: e - ahimè! - il primo passo possibile è l'Italia. Avevamo fermato completamente quel tipo di immigrazione. non ripeto la preoccupazione che abbiamo manifestato qualche giorno fa rispetto al fatto che vi sono alcune fabbriche italiane o con partecipazioni di Agusta-Westland e di Finmeccanica che - ahimè - producono armi in quel Paese. Vorremmo essere rassicurati che non finiscano in mani

L'Europa, prima delle banche, dovrebbe pensare a difendere i propri cittadini, secondo il modesto parere della Lega Nord. Altrimenti,

vorremmo sperare per il meglio, ma le vogliamo esternare la nostra preoccupazione: prepariamoci anche al peggio!

ha ripetuto poco fa anche qui, in Senato, che di fronte a quello che sta accadendo in Libia, di fronte all'orrore di un dittatore disperato che bombarda il suo stesso popolo mietendo centinaia di vittime e in un crescendo paranoico sogna di trascinare la Libia e il mondo intero nel suo destino di morte, la misura è colma: ogni limite è stato oltrepassato e a questo punto - uso le sue parole - non possiamo non levare la nostra voce. Mi faccia dire, signor Ministro, che era ora. Finalmente! Accogliamo le sue parole con sincero sollievo perché segnano un punto di svolta nella linea tenuta fin qui dal Governo: una linea sbagliata che non solo ci ha impedito di capire cosa stava accadendo nel nostro cortile di casa, nel Mediterraneo, ma ci ha anche portato - questa è la dura verità - sulla soglia di un vero e proprio isolamento internazionale. Signor Ministro, parlo di un isolamento politico e perfino morale, una condizione che non avevamo mai conosciuto nella storia della Repubblica. In questo caso, non c'entra niente la politica di buon vicinato con la Libia, che certamente ha rappresentato un elemento di continuità della nostra politica estera. Come ebbe a dire tante volte il presidente Andreotti, gli amici si possono scegliere, i vicini no. E la Libia è un nostro vicino con il quale, se non vogliamo fare la guerra, dobbiamo fare la pace. Ma un conto è il buon vicinato, un altro conto è l'umiliante esaltazione di un dittatore. Un conto è il realismo politico, quello stesso realismo politico che ci ha portato a realizzare il Trattato di amicizia con un Paese vicino, un altro conto è indicare la Libia di Gheddafi come modello per il mondo arabo, come lei ha fatto poco più di un mese fa, signor Ministro, a Governo tunisino già caduto, in piena crisi nel Mediterraneo, in una sconcertante intervista al «Corriere della Sera». Aver tenuto caparbiamente quella linea indifendibile, la linea che in tutto il mondo è diventata del "*do not disturb*", del "non disturbiamo" Gheddafi, ha nuociuto gravemente alla credibilità dell'Italia. Su quella linea siamo stati messi in minoranza in Europa nelle stesse ore nelle quali il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e la stessa Lega araba, come lei ha ricordato, pronunciavano parole di condanna durissima nei confronti del regime libico e invocavano la responsabilità di proteggere le popolazioni intimando il pieno rispetto del diritto delle genti. Ora quella linea è stata abbandonata dobbiamo voltare pagina per affrontare con serietà e responsabilità, ciascuno nel proprio ruolo, ma insieme, le sfide del presente e del futuro. In primo luogo, le sfide del presente, che assumono le vesti di una drammatica crisi di emergenza, sul piano umanitario, innanzitutto.

il problema di migliaia di libici che in questo momento vivono una condizione drammatica, sotto il fuoco dello stesso Esercito del loro Paese, al comando di un dittatore che non si fa scrupolo di colpire la sua stessa popolazione. C'è un'emergenza energetica, che potrebbe interessare il nostro Paese. C'è indubbiamente un'emergenza economica. C'è soprattutto il tema di un'accoglienza e di un soccorso a profughi e rifugiati. Profughi e rifugiati, signor Ministro, non immigrati. È una fattispecie profondamente diversa quella con la quale avremo a che fare nelle prossime settimane e mesi. Noi condividiamo, signor Ministro, la sua proposta di confrontare idee e proposte per la gestione dell'emergenza in Parlamento, perché questa è la sede naturale nella quale maggioranza e opposizione si confrontano e collaborano nell'interesse del Paese, utilizzando a tal fine le Commissioni affari esteri e diritti umani. Chiediamo tuttavia di discutere in modo ampio e approfondito le linee di azione di questa gestione dell'emergenza in un dibattito su una relazione del Presidente del Consiglio, proprio perché questi temi hanno a che fare con la collegialità delle responsabilità del Governo. Vogliamo essere chiari, signor Ministro: tanto più le proposte che ascolteremo saranno di svolta rispetto alla conduzione recente, per esempio in tema di immigrazione, tanto più noi potremo dare il nostro contributo e il nostro apporto ad una gestione

noi non abbiamo condiviso, lo abbiamo detto tante volte in quest'Aula, il modo con cui è stato gestito il problema dell'immigrazione nel rapporto bilaterale con la Libia, peraltro ben al di là e ben oltre i termini affrontati nel Trattato di amicizia italo-libico. Con alcune norme introdotte negli scorsi mesi è stato dato un sostanziale appalto bilaterale alla Libia nella gestione della partita immigrazione, esautorando completamente qualunque ruolo dell'Europa e perfino dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, che ha il ruolo istituzionale di presiedere a una funzione tanto delicata di sorveglianza su un tema così decisivo. Su questi temi vogliamo un confronto stringente, purché sia serio e trasparente. Vi è poi il tema di fondo, della prospettiva, del futuro. Concludo, signora Presidente, con una battuta su questo: siamo nel pieno di una svolta storica nel Mediterraneo. Come tutte le svolte storiche - ce lo siamo detti già altre volte possono esserci sbocchi positivi, e possono esserci degli sbocchi preoccupanti e negativi. Dobbiamo lavorare e fare tutto quanto è possibile, come italiani e come europei, questa svolta esprima al meglio tutte le sue potenzialità, perché davvero possiamo trovarci in presenza di un'evoluzione positiva del mondo arabo verso la democrazia e lo sviluppo. Ci sono dei valori fondamentali da tutelare in questo delicato passaggio: c'è il valore della libertà dei popoli, c'è il valore della democrazia, c'è, ad esempio, il valore della sicurezza e dell'esistenza dello Stato d'Israele (vediamo in questi giorni, con la vicenda delle navi iraniane, quanto questo valore possa essere messo in discussione). Tutto questo chiede una politica estera nuova: quella politica estera per l'Italia alla quale noi siamo pronti a dare tutto il nostro contributo. Signora Presidente, signor Ministro, desidero esprimerle sostegno e soddisfazione per la relazione che ha voluto comunicarci in riferimento ai gravi e tragici fatti che si stanno determinando in Libia. Speravo, come molti di noi probabilmente, che un tema così importante in un momento così difficile avesse suggerito un po' a tutti di seguire quella linea comune tale da evitare polemiche e possibili recriminazioni o addirittura atteggiamenti colpevoli. Del resto, è molto complesso immaginare che qualcuno potesse aver avuto cognizione di quanto stava accadendo in modo preciso nella sponda meridionale del Mediterraneo: in Tunisia, in Egitto, e in modo particolare in Libia. Oggi però ho ascoltato degli interventi che effettivamente non vanno in quel senso. Sono rammaricato che il collega Tonini abbia voluto sottolineare una specie di palese e straordinaria contraddizione sulle posizioni del Governo e anche in riferimento alla relazione del Ministro. collega Tonini, indubbiamente non è un pregio per molti, e purtroppo tra questi molti rientrano anche autorevoli esponenti del Partito Democratico.

collega Latorre quando è intervenuto in dichiarazione di voto in riferimento proprio ai rapporti tra Italia e Libia, al Trattato. Dice il collega Latorre: «Dunque noi voteremo a favore di questo Trattato. Un rinvio - vedete - oggi suonerebbe come un incomprensibile atto di ostilità nei confronti di quel Paese. Si può consolidare un quadro di relazioni, non solo di partenariato energetico, ma anche per le nuove opportunità di mercato che si aprono per il nostro Paese e pure sul piano culturale. Non vorrei che si dimenticasse che la Libia è l'unico Paese arabo in cui si parla italiano. Un riscatto storico, dunque, una utile e lungimirante operazione diplomatica» - stiamo parlando del Trattato «verso il mondo arabo. Un Trattato che corrisponde agli interessi generali dell'Italia e che dunque, con questa impostazione, noi sosterremo con il nostro voto». É passato circa un anno da questa dichiarazione, ma ve ne sono anche di più recenti.

è una forte stanchezza del suo regime, ma che certamente Gheddafi ha ancora un rapporto solido con una parte della società libica e che la crisi economica lì non aveva colpito come in altri Paesi.

nei suoi incontri con Gheddafi avesse parlato mai di diritti umani, risponde: «In modo diretto, no. Se ne accennava, a volte, ma non si metteva niente all'ordine del giorno...».

della Sera», dove si legge che «Ora, naturalmente, nessun Governo europeo può astenersi dal condannare le violente repressioni di Bengasi e di Tripoli. Noi, in particolare, abbiamo il diritto e il dovere di alzare la voce contro Gheddafi e i suoi metodi. Ma cerchiamo almeno di farlo senza cogliere l'occasione per combattere una ennesima battaglia di politica interna. Nel momento in cui in Libia si muore lo spettacolo sarebbe particolarmente indecoroso». Vorrei concludere, signora Presidente,

presidente della Commissione europea Barroso, che, dopo un incontro con l'Alto commissario dell'ONU per i diritti umani, affronta il tema della possibilità di migrazioni dal Nord Africa affermando dobbiamo rispondere al problema in modo europeo. Noi ce lo auguriamo, presidente Barroso, perché sicuramente questo non può essere un problema italiano, ma deve essere un problema europeo. Grazie ancora, signor Ministro, e grazie per l'attività che state svolgendo.

il disegno di legge in esame, avente ad oggetto la disciplina del processo produttivo e di commercializzazione relativa ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, proviene dalla Camera dei deputati, al termine di un *iter* che ha portato all'approvazione di un testo condiviso dalle diverse forze politiche, frutto di un lavoro concordato e *bipartisan*. Tale accordo unanime si è manifestato nella condivisione delle finalità del testo e nelle modifiche apportate rispetto alle iniziative originarie, anche a seguito di una serie di audizioni dei diversi soggetti e categorie interessati. Oggetto fondamentale del provvedimento, secondo quanto accennato, è il settore dei prodotti ortofrutticoli, definiti comunemente di quarta gamma, che vengono preselezionati, mondati, lavati e confezionati pronti per il consumo. Si tratta di prodotti che possono acquisire ulteriore valorizzazione in relazione alle caratteristiche del prodotto di base, quali a titolo esemplificativo la provenienza geografica o la coltivazione biologica, o al confezionamento delle miscele. I prodotti in questione sono presenti nel mercato non soltanto tramite le catene della grande distribuzione organizzata, ma anche attraverso i servizi di ristorazione e le mense scolastiche, ed è un profilo tenuto in particolare considerazione sia nell'ispirare sia nel definire il testo in esame. In base a quanto premesso, occorre pertanto rilevare che la disciplina proposta risponde in primo luogo alla necessità di fornire la migliore normativa nei confronti di un settore che appare oggettivamente in forte crescita, soprattutto alla luce delle tendenze al consumo degli ultimi anni, nel corso dei quali il mercato dei prodotti di quarta gamma, configurabile inizialmente in un ambito di nicchia, è stato oggetto di una espansione che ormai giustifica il superamento di tale considerazione. In questo senso, occorre altresì rilevare che l'evidente crescita del settore ha subito un rallentamento nell'ultimo periodo, legato probabilmente a un ancora diffuso margine di scetticismo e diffidenza, in ragione sia di motivazioni di carattere economico, soprattutto con riferimento ai prezzi più elevati rispetto agli ortofrutticoli freschi, sia di una ancora radicata preferenza per le verdure fresche e i consumi tradizionali, collegata forse anche alla maggiore deperibilità dei prodotti di quarta gamma. quanto appena ricordato, appare evidente l'opportunità di predisporre una nuova ed efficace normativa nei confronti di un settore che tuttora dimostra grandi potenzialità di sviluppo, soprattutto se inserito in un contesto di crisi del complessivo comparto agroalimentare. Nell'ambito della disciplina proposta occorre richiamare l'attenzione sulle finalità che hanno ispirato il disegno di legge, costituendone il nucleo centrale, ovvero l'esigenza di garantire sia la qualità alimentare e nutrizionale del prodotto, sia la sicurezza dello stesso, in relazione ai requisiti igienico-sanitari, sia l'informazione e la tutela del consumatore in particolare. I profili ora richiamati possono essere definiti come i principi generali della disciplina proposta, contenuti essenzialmente negli articoli 3 e 4 della stessa. Gli articoli 1 e 2, in stretta correlazione, sono volti a individuare l'oggetto del provvedimento e la definizione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, con particolare riferimento alle diverse fasi del processo produttivo di lavorazione, tutte in ogni caso finalizzate alla valorizzazione del prodotto. Gli articoli 3 e 4, secondo quanto anticipato, dettano le disposizioni di maggior contenuto, riferite alle procedure di commercializzazione e alle disposizioni di attuazione della disciplina. In particolare, l'articolo 3 stabilisce i criteri generali concernenti le due fasi del confezionamento (comma 1) e della distribuzione (comma 2). Appare opportuno rilevare che i prodotti in questione possono essere confezionati singolarmente o in miscela, restando peraltro consentita una limitata aggiunta di ingredienti di origine vegetale non freschi o secchi, secondo una percentuale fissata dal decreto ministeriale di cui al successivo articolo. Quanto alla distribuzione, essa può avvenire lungo l'intera filiera o tramite distributori automatici, nel rispetto dei parametri stabiliti dal decreto ministeriale citato. L'articolo 4 prevede per l'attuazione della disciplina l'emanazione di un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, con il quale sono definiti, in linea con la normativa comunitaria, i parametri igienico-sanitari delle diverse fasi del processo produttivo e i requisiti qualitativi minimi, nonché le informazioni obbligatorie a tutela del consumatore che devono risultare sulle confezioni.

il mercato dei prodotti di quarta gamma (ovvero di quei prodotti agricoli rappresentati quasi esclusivamente da ortaggi e frutta distribuiti già preconfezionati o imbustati) negli ultimi dieci anni è fortemente aumentato: in Italia, il fatturato di questi prodotti è considerevolmente cresciuto, tanto da far diventare il mercato italiano il secondo in Europa. Questi prodotti, pronti al consumo, rispondono al bisogno del consumatore di ridurre i tempi di preparazione, ma anche di eliminare - o per lo meno ridurre - il volume degli scarti di cucina. Per questo motivo, è sorta la necessità di adottare una legge che disciplini la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma destinati all'alimentazione umana. Bisogna tuttavia considerare che i consumatori hanno ancora un certo scetticismo nei confronti dei prodotti di quarta gamma. Infatti, l'evidente crescita del settore ha subito un rallentamento nell'ultimo periodo, legato probabilmente ad un ancora diffuso margine di diffidenza dei consumatori stessi, in ragione sia di motivazioni di carattere economico (soprattutto con riferimento ai prezzi, che sono molto più elevati rispetto ai prodotti ortofrutticoli freschi), sia di una ancora radicata preferenza per le verdure fresche e i consumi tradizionali, collegata, in parte, alla convinzione di una loro maggiore genuinità e, in parte, anche alla maggiore deperibilità dei prodotti di quarta gamma. Dunque, non tutti apprezzano i vantaggi dei prodotti di quarta gamma. Si tratta di persone che hanno preferenze verso consumi più tradizionali e che non hanno l'abitudine di utilizzare e di consumare questi prodotti innovativi. Ci sono - quindi - anche gli scettici e i diffidenti. C'è chi lamenta che questi prodotti non siano più o meno buoni o genuini, ma soprattutto i consumatori si lamentano per i prezzi, che sono senz'altro più elevati rispetto a quelli delle verdure fresche. È, soprattutto, il processo di produzione (che va dalla coltivazione alla distribuzione refrigerata) che ha un costo elevato e, proprio per questo motivo, i prodotti di quarta gamma costano di più di quelli freschi. Le insalate e le verdure di quarta gamma sono più deperibili degli equivalenti prodotti di prima gamma, e il punto debole è individuato, in base ai giudizi dei consumatori, soprattutto in riferimento alla carica batterica a causa della quale le verdure di quarta gamma sarebbero incriminate. Altro argomento controverso riguarderebbe i principi nutritivi di detti prodotti, in quanto sono in molti a pensare che vadano persi in seguito ai trattamenti subiti dai prodotti stessi. Certamente, durante il taglio e il lavaggio si verifica una certa perdita di vitamine, ma senz'altro ciò succede anche a casa quando si compiono le stesse operazioni sui prodotti freschi. Le verdure di quarta gamma, quindi, hanno una vita molto più breve dell'equivalente fresco, per cui alla fine è probabile - e questo, magari, giustifica un po' chi utilizza questi prodotti - che di sostanze nutritive, quali vitamine, ce ne siano di più. Questi sono i pro e i contro, ma è certo che oggi il consumo di questi prodotti di quarta gamma raggiunge il fatturato di spesa della stessa pasta: ciò vuol dire che i consumatori italiani, in maggioranza, preferiscono utilizzarli. Ecco, quindi, il motivo del provvedimento al nostro esame, nato per garantire la sicurezza e la qualità alimentare anche di questi prodotti, visto l'uso crescente che gli stessi consumatori italiani ne fanno. È fondamentale, dunque, evitare il rischio di frodi e l'utilizzo di prodotti di origine poco certa e garantire al consumatore la qualità della materia all'origine. Si tratta sempre del solito discorso della tracciabilità, che, comunque, riguarda tutti i prodotti alimentari che provengono dalla terra. È necessario, nel contempo, garantire sia la qualità nutrizionale del prodotto, sia i requisiti igienici. Il testo unificato approvato dalla Commissione agricoltura regolamenta questo prodotto, garantendo soprattutto - e principalmente - il consumatore. Il testo uscito dalla Commissione agricoltura del Senato rappresenta, a nostro avviso, un provvedimento ben fatto, che definisce correttamente i prodotti di quarta gamma, di cui non solo sottolinea le buone pratiche di lavorazione (come la selezione, la cernita, la monda, il taglio, il lavaggio, l'asciugatura e il confezionamento in busta o nella vaschetta sigillata), ma regola anche la commercializzazione. A nostro avviso, è importante la precisazione che, nell'eventualità in cui il prodotto venga destinato alle scuole, le produzioni vegetali utilizzate provengano prevalentemente dal territorio nazionale e ne venga garantita quindi la tracciabilità. Nel corso dell'*iter* del provvedimento, sia alla Camera che al Senato, si è giunti all'approvazione di un testo ampiamente condiviso da tutte le parti politiche. Di conseguenza, c'è stata una voce unanime, siamo stati tutti d'accordo e abbiamo concordato le modifiche apportate al testo unificato. In particolare, presso la Commissione agricoltura del Senato, su parere favorevole del relatore, sono state accolte due modifiche al testo trasmessoci dalla Camera, presentate dai colleghi del Gruppo del Partito Democratico, volte principalmente ad introdurre, attraverso un apposito decreto ministeriale, l'obbligo di utilizzare imballaggi biodegradabili, precisando che tale misura dovrà essere adottata secondo moduli graduali e progressivi, in modo tale da non creare problemi agli operatori del settore. onorevole relatore, onorevole rappresentante del Governo, mi sia consentito esprimere una grande perplessità non tanto sul merito del provvedimento, quanto piuttosto sul metodo di lavoro seguito dalla maggioranza: infatti, nell'esprimere il nostro giudizio favorevole nei confronti dei contenuti del provvedimento in esame, non posso non evidenziare il poco chiaro, se non addirittura poco corretto, comportamento del relatore, il quale, prima, nel corso dell'*iter* in Commissione, accoglie delle giuste modifiche e integrazioni al testo e successivamente, in quest'Aula, ne chiede la soppressione, proponendo con emendamento l'esatto contrario di quanto deciso in Commissione.

già dagli interventi che mi hanno preceduto e dalla relazione del senatore Sanciu si comprende di cosa stiamo parlando ma secondo me vale la pena dare chiarezza e

Si tratta, di fatto, di prodotti freschi, che vengono selezionati, lavati e poi confezionati confezionati e che siamo già da un po' abituati a trovare sugli scaffali, sia della grande distribuzione che del piccolo dettaglio, come pure nei distributori. Si presentano come prodotti non troppo significativi dal punto di vista quantitativo, ma in realtà rappresentano un segmento di mercato con delle grandi potenzialità e un elevato contenuto di innovazione, le cui dimensioni reali sono già state descritte nell'intervento del senatore Di Nardo. La qualità dei prodotti, la sicurezza degli stessi, la tracciabilità dell'origine pongono oggi a carico dell'impresa agricola e agroalimentare delle richieste inedite, e creano una inedita connessione tra produttori e consumatori. Questo fatto assegna alla politica e alle istituzioni, ciascuno nell'ambito delle specifiche competenze, il compito di concorrere alla costruzione di un nuovo patto tra chi produce e chi consuma. Il consumatore è sempre più attento, sempre più forte, e quindi è in grado anche di condizionare le scelte produttive. Ciò è tanto più forte nel nostro Paese, ove la cultura del "cibo buono e sano" modella le nostre abitudini alimentari e promuove in modo deciso la qualità delle produzioni. Per i produttori, quindi, la qualità del prodotto, la sua autenticità, la sua riconoscibilità offrono scenari di sviluppo importanti, e a volte inediti, che richiedono però capacità di innovazione, disponibilità all'investimento e tempi lunghi di programmazione. Diventa così necessario definire le regole, certe e precise, su cui fondare il nuovo patto tra il consumatore e il produttore, che diventano la garanzia di riferimento per entrambi. In questo scenario, i prodotti di quarta gamma si collocano a pieno titolo, e questo provvedimento, insieme ai decreti ministeriali che seguiranno, contiene queste regole di garanzia. In particolare, la definizione di prodotto fresco riferito ad un prodotto che si presenta come confezionato richiede condizioni precise di trattamento igienico-sanitario per la sicurezza di salubrità del prodotto; come pure sono importanti le disposizioni, già contenute nella proposta di legge, che impongono l'indicazione dell'origine e del contenuto della confezione: in questo modo, noi veniamo anche a rafforzare ancora una volta il convincimento che per i nostri prodotti la tracciabilità è una condizione indispensabile per la costruzione di un mercato di leale concorrenza. Il testo che quest'Aula si prepara a votare va sicuramente in questa direzione ed è il frutto di un lavoro congiunto delle forze politiche, che ne é garanzia di longevità. Per questo motivo, vale la pena di valutarne la completezza, come abbiamo fatto in Commissione agricoltura. In quella sede, infatti, è emerso un aspetto molto rilevante che il testo uscito dalla Camera non aveva affrontato, ossia il tema dello smaltimento degli imballaggi, che va visto alla luce sia degli obiettivi di sostenibilità ambientale che ci vengono assegnati, sia della crescente onerosità che il ciclo di smaltimento dei rifiuti determina oggi. All'inizio di quest'anno, è infatti diventato obbligatorio per le imprese della distribuzione l'utilizzo di buste biodegradabili, e non possiamo pensare di di approcciarci oggi ad una legislazione che determina sicuramente un aggravio nell'utilizzo dei materiali da imballaggio senza porci il tema del costo ambientale ed economico del loro smaltimento. In Commissione il Partito Democratico ha presentato due emendamenti, condivisi dall'intera Commissione, che andavano a correggere questo aspetto, prevedere un prevedere un decreto ministeriale che stabilisse l'obbligo di utilizzo di imballaggi biodegradabili, avendo cura ovviamente di tener tener conto delle ragioni degli operatori, e quindi della gradualità dell'applicazione. Purtroppo, apprendiamo in queste ore che sono stati presentati in Aula due emendamenti da parte della maggioranza che di fatto riportano al contenuto del testo approvato alla Camera. Si decide, quindi, consapevolmente di giungere all'approvazione di un provvedimento che è senz'altro incompleto e che richiederà un successivo provvedimento, così com'è successo nel caso delle buste che ho appena ricordato. Credo valga la pena di utilizzare l'unico aspetto positivo del bicameralismo del nostro ordinamento, che, se da un lato allunga i tempi, dall'altro consente di addivenire alla correzione*in itinere*,

per arrivare all'approvazione di un provvedimento moderno su cui non sia necessario intervenire il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

non serve nessuna replica. Dico solo che c'è un confronto anche con l'opposizione per trovare la sintesi su due emendamenti che il relatore ha già depositato. Per quanto riguarda l'emendamento all'articolo 2 c'è già una condivisione; per quanto riguarda l'emendamento all'articolo 4 abbiamo concertato un testo.

1a Commissione permanente, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nel presupposto che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie "tutela della salute" e "alimentazione" che, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono attribuite alla competenza concorrente, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, considerando che gli articoli 1, 2 e 3 contengono disposizioni di principio e che, all'articolo 4, è opportunamente prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per l'adozione dei decreti ministeriali di attuazione. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

L'emendamento 2.100 si rende necessario perché i prodotti di quarta gamma necessitano di un confezionamento in atmosfera protettiva per evitare ossidazioni o degradazioni che ne pregiudichino la salubrità o l'idoneità al consumo. Allo stato attuale della scienza, tuttavia, i polimeri utilizzabili per gli imballaggi biodegradabili risultano permeabili al vapore acqueo e pertanto non assicurano la corretta conservazione dei prodotti stessi, che andrebbero a deperire in tempi rapidi, nonostante il mantenimento di idonee temperature di conservazione lungo la catena di produzione e commercializzazione. comma 1, sostituire le parole: «contenitori sigillati» con le seguenti: «vaschette sigillate».

Gruppo dell'Italia dei Valori, vista anche la risposta che abbiamo avuto dal relatore, voterà a favore del provvedimento

Presidente, a nome del Gruppo della Lega Nord, non posso che unirmi alle dichiarazioni dei colleghi che mi hanno preceduto su questo provvedimento, che sicuramente è importante e va nella direzione della trasparenza nei confronti di

la collega Bertuzzi ha evidenziato l'importanza di questo settore. Abbiamo condiviso sin dall'inizio questo provvedimento. Del resto, abbiamo contribuito con un emendamento per accrescere la qualità sia dei prodotti che dell'imballaggio. ringraziare il relatore e il presidente Scarpa Bonazza Buora perché hanno ritirato un emendamento che andava a cancellare questa modifica, spinti da preoccupazioni anche comprensibili che riguardavano la sicurezza alimentare e i costi eccessivi, nonché la carenza di materia prima. Non solo siamo certi che non vi sono problemi rispetto ai problemi di conservazione (lo dicono le esperienze testate dai laboratori universitari, dalle imprese che già producono questo materiale), crediamo anche che proprio nei materiali ecocompatibili, biodegradabili stia la nuova frontiera per la competitività delle nostre imprese. Qui stiamo facendo un servizio sia ai consumatori che al futuro

molta gente che lavora in questo settore, in forte espansione nel comparto agroalimentare del nostro Paese. Mi rallegro che ancora una volta abbiamo potuto registrare, anche alla luce degli ultimi interventi del senatore Di Nardo del senatore Di Nardo e della senatrice Pignedoli, una comunanza di vedute, una capacità di armonizzazione di pensiero fra tutti i senatori che si occupano quotidianamente di problematiche agricole e che lavorano nella Commissione che ho l'onore e il piacere di presiedere: di questo non posso che rallegrarmi. È una conferma di una capacità di stare insieme, di lavorare nell'interesse dell'agricoltura che la Commissione agricoltura del Senato ogni giorno realizza.

14.000 ettari in Sardegna, dove insiste un poligono militare, il poligono sperimentale di addestramento interforze. In questo In questo territorio così sconfinato e di incomparabile bellezza (un territorio che noi Sardi vorremmo venisse utilizzato per altri scopi, e non già per questo asservimento

sia italiane che straniere; vi operano il Centro italiano di ricerche aerospaziali dell'università di Roma, l'Agenzia spaziale europea e, così ci viene detto, anche numerose ditte straniere che producono armi. armi. Il motivo di questa mozione è che il Gruppo del Partito Democratico, nella sua interezza, ritiene di dover impegnare il Governo in un'azione di chiarificazione che nel corso degli ultimi dieci anni non si è realizzata. Il problema è il seguente: si ha motivo di ritenere che l'utilizzo di armi, di proiettili e comunque di materiali che fanno parte del sistema di addestramento e di sperimentazione possa aver provocato una serie di patologie di notevole gravità. Si parla di possibili tumori, al sistema linfatico in particolare, che potrebbero aver colpito gli uomini e gli animali. È necessario fare chiarezza e verificare se esista o meno il cosiddetto nesso di causalità fra l'utilizzo di questi materiali, di queste armi e di questi esplosivi, e la presenza, che appare superiore alla media, delle patologie cui ho fatto cenno.

L'unica indagine epidemiologica finora svolta è stata definita descrittiva. Si sono, cioè, praticamente contati i casi o di malattie contratte o di decessi, senza aver potuto acclarare, con quella che viene definita indagine epidemiologica *ad hoc*, se effettivamente sussistano o meno le ragioni di causalità che ancora non sono state inequivocabilmente dimostrate. Debbo dire, signor Presidente e colleghi, che il testo di questa mozione è stato integrato e corretto grazie all'impegno dei colleghi che operano nella Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uranio impoverito, in particolare del suo presidente Costa, ma anche del collega Gamba e degli altri firmatari di una mozione analoga.

siamo pervenuti a dei testi che potremmo definire concordati. Il risultato che finalmente ci proponiamo di ottenere è che dopo molte dopo molte Commissioni che hanno operato negli anni passati, dopo migliaia di articoli che sono stati scritti, dopo tutta una ridda di ipotesi

rilevando l'eventualità che possano essere stati commessi reati di omicidio plurimo, omissione di atti d'ufficio e inquinamento ambientale. Il dispositivo, signor Presidente e colleghi, cercherò di riproporlo in maniera sintetica. Entro il 30 giugno 2011 il Governo si impegna a portare a termine l'analisi da parte della commissione tecnica di esperti; lo stesso Governo si impegna entro il dicembre 2011: « a concorrere efficacemente, per quanto di competenza, all'avvio di un'indagine sanitaria ed epidemiologica tendente ad accertare natura, entità, incidenza e prevalenza delle patologie tumorali e malformative e della mortalità, individuandone le determinanti causali, anche tramite l'affidamento all'Istituto superiore di sanità dell'incarico di costituire un *board* scientifico».

Mi riferisco all'eventuale sospensione delle attività del poligono interforze, ove dall'analisi dei dati raccolti da parte della commissione tecnica di esperti, ovvero da ulteriori indagini disposte anche con il concorso della Regione sarda, dovessero emergere oggettive situazioni di rischio per gli abitanti delle aree vicine al poligono e per il personale della Difesa. Questa richiesta, che avanziamo avendola avendola concordata per le vie informali con i colleghi del Governo e della maggioranza cui ho fatto cenno poco fa, costituisce una straordinaria novità, perché definisce in termini espliciti la sensibilità, oltre che del Governo, anche delle Forze armate rispetto a una materia che pretende il riconoscimento del primato della salute delle persone rispetto ad ogni altra esigenza, ancorché di valore internazionale. Si impegna infine il Governo ad assicurare un costante monitoraggio delle condizioni ambientali dell'area, rendendo possibile l'accesso ai relativi dati sia alle amministrazioni locali che alle associazioni interessate, al fine di garantire che il prosieguo dell'attività del poligono avvenga in totale sicurezza. Sinteticamente potremmo dire che verrà squarciato il velo di una forma di reticenza o di ritrosia ad andare nel profondo delle cose, e riteniamo, se questa mozione verrà approvata di capire), di poter ottenere finalmente dal nostro Governo e dalla Regione sarda quelle risposte serie, efficaci e puntuali che finora - purtroppo - sono mancate.

presentare una mozione relativamente al problema che è stato sollevato e indicato nella mozione di cui è primo firmatario il collega Scanu. Si tratta della vicenda relativa all'attività di uno dei più importanti poligoni sperimentali attualmente in esercizio: mi riferisco anche detto di Salto di Quirra, attesa la grande ampiezza territoriale che questo dispiega. Esso è utilizzato per la sperimentazione di ogni tipologia di armamento

tende a mettere in relazione alcune incidenze di patologie, che sarebbero state riscontrate negli abitanti delle zone finitime all'estensione del poligono, con le attività e svolte nell'ambito del poligono stesso. Ciò ha comprensibilmente suscitato un allarme e delle preoccupazioni.

del poligono per verificare la presenza di eventuali sostanze inquinanti sia aerodisperse, sia nel suolo, nelle acque o negli animali. Inoltre, tale attività di caratterizzazione è stata assegnata mediante una procedura di evidenza pubblica a società indipendenti e qualificate le cui attività, quindi, sono estranee di per sé all'Amministrazione della difesa, e dovrebbero quindi fornire maggiori garanzie di trasparenza e attendibilità rispetto alle preoccupazioni che lamentava e ricordava anche il collega Scanu.

se non durante lo svolgimento delle attività di sperimentazione, che sono poi autorizzate e concordate nell'ambito del Comitato paritetico che,

da un'approfondita analisi dell'impatto ambientale, volta proprio a garantire la salvaguardia della popolazione e la tutela dell'ambiente, oltre che della sicurezza del personale stesso che partecipa a tali attività di sperimentazione militare.

i Gruppi del PdL e della Lega Nord convengono sicuramente sulla necessità di svolgere in massima trasparenza le attività di verifica e di accertamento

di accertamenti sanitari ha iniziato e si prefigge di continuare a svolgere - e sul fatto che, nel caso in cui questi accertamenti, come noi non crediamo, dovessero portare al riscontro di effettivi rischi per la popolazione, oltre che per il personale stesso della Difesa che partecipa a a questo genere di attività, si debbano sospendere le attività addestrative e sperimentali presso il poligono di Salto di Quirra, prendendo ovviamente in considerazione i necessari provvedimenti alternativi. Poiché è evidente che si deve dare una risposta in termini di assoluta certezza e trasparenza a queste preoccupazioni, senza arrivare a conclusioni precostituite, che in

di massima trasparenza riguardo all'effettiva mancanza di rischi per le popolazioni e per gli operatori della Difesa.

condivisione dell'obiettivo, che non può che essere quello di garantire il massimo della tutela della salute per tutte le persone coinvolte, vale a dire gli abitanti che vivono nelle zone confinanti e naturalmente gli operatori militari dell'Amministrazione della difesa che in prima persona sono coinvolti, senza dimenticare però che in questa vicenda devono anche essere preservati e ricordati gli aspetti occupazionali, che trovano un forte legame con le attività svolte in quel territorio e che non a caso costituiscono invece oggetto di preoccupazione proprio da parte di alcune amministrazioni ed enti locali della zona, oltre che evidentemente degli stessi operatori della Difesa. Crediamo che attraverso questo confronto si possa arrivare ad impegni comuni. Ovviamente ascolteremo quanto ci dirà in merito il rappresentante del Governo, onorevole Cossiga, siamo certi che si possa, pur con il confronto tra le due mozioni, arrivare al raggiungimento di quell'obiettivo comune che mi sembra condiviso, al di là delle premesse e delle posizioni di partenza rispetto a questa vicenda.

che entrambe le mozioni (ma, permettetemi di dire, in maniera molto più chiara quella presentata dal Partito Democratico a prima firma del senatore Scanu) affrontano un tema che è scabroso ai giorni nostri, quando le tecnologie sono applicate alle pratiche e all'arte della guerra, con esempi che dalla guerra in Iraq si portano sino all'esperienza nell'Europa occidentale e, purtroppo, nelle guerra sporche che si combattono un po' in tutto il mondo. È il tema del rapporto tra queste tecnologie e la capacità offensiva delle armi, anche al di là dell'intenzione di chi le usa contro il nemico e l'avversario, perché

Credo che l'approccio di queste mozioni sia moderno, perché è l'opposto del sensazionalismo ed è la presa d'atto che l'allarmismo lo crea l'indifferenza e la scarsa trasparenza; non la ricerca di evidenze scientifiche, non l'applicazione delle migliori tecniche d'indagine, non quindi la cura che gli Stati democratici pongono nel tenere indenni i propri eserciti e le proprie popolazioni dall'uso improprio delle tecnologie di guerra. Sono altri due i punti che le mozioni in qualche modo evocano. Il primo è quello di una concentrazione, secondo me impropria e in contrasto anche con quanto prevede la legge n. 104 del 1990,

(ce ne sono altre che vedono una concentrazione impropria di servitù militari) per come si è dispiegata la storia e l'assetto delle Forze armate di pace in Italia,

C'è già stata nei giorni scorsi alla Camera dei deputati una prima risposta che ci dà la dimensione e l'urgenza delle cose che la mozione

delle richieste di indennizzo che oggi gravano sull'amministrazione dello Stato da parte del personale militare, il 15 per cento proviene da quel poligono: sono 68 le richieste di indennizzo, tutte per tumori,

come non sia stata casuale la sua istituzione. Evidentemente, *ad adiuvandum* rispetto all'attività del Governo, si è voluto che il Parlamento avesse un periscopio su questo argomento che tanto interessa gli italiani, civili e militari, e non soltanto gli italiani. Devo dare atto in via estemporanea, dal momento che, evidentemente, la Commissione, nei tempi e nei modi dovuti, renderà la sua relazione conclusiva, che si sta lavorando con molta passione e con unanime consenso. Ogni qualvolta si adottano determinazioni non c'è maggioranza e minoranza, tanta è la condivisione dell'interesse comune e pubblico

Noi auspichiamo, perché questa era l'intenzione dei presentatori, che sia la prima che la seconda mozione siano votate da maggioranza e opposizione, dando così all'esterno, a chi ci ascolta, a chi è interessato, a chi soffre e a chi ha la preoccupazione - mai sia! - di dover soffrire, che il Parlamento è tutto intero dalla parte della verità, e più segnatamente dalla parte dei militari in missione di pace e dei civili che li seguono e collaborano

su questa mozione perché si tratta di una questione molto delicata e grave, che non trae origine da accertamenti e da segnalazioni verificatisi solo in tempi recenti. Infatti sono anni che si parla di questa situazione. Ci sono state delle indagini scientifiche epidemiologiche alle quali ho anche partecipato nel 2005 prima di entrare in quest'Aula

Questi accertamenti avevano segnalato una situazione nelle popolazioni residenti all'interno della Sardegna piuttosto gravi, con particolare riferimento ad alcune aree che sono quelle industriali e minerarie.

venivano segnalati degli eccessi di malattie tumorali in capo alla popolazione che abitava all'interno dei Comuni

nel tempo e quindi di segnalare i fattori e le situazioni di rischio e di intervenire in maniera più consona e proficua. A ciò ci richiama il tanto noto principio di precauzione che sarebbe opportuno concretizzare, partendo da questo fenomeno specifico.

con un'intera comunità, che - come è stato detto, da ultimo dal collega Casson - non da oggi e non da poco tempo è molto preoccupata per le condizioni

discussione. Riteniamo che il dato per cui il Senato impegnerà il Governo - approvando, mi auguro, all'unanimità entrambe le mozioni che stiamo discutendo, con l'accordo con l'accordo del Governo stesso - sia più importante e prevalente rispetto a qualsiasi altra cosa, perché forse diamo risposta alle preoccupazioni di quella comunità, avremo quello studio epidemiologico che dovrà darci risposte definitive in relazione ad una situazione che è gravissima.

Vorrei però fosse chiaro, soprattutto alla comunità di quel territorio, che ciò non significa una diminuzione dell'attenzione da parte nostra su quello che sta avvenendo.

sopralluogo sul posto. Noi non siamo in grado di rinviare ulteriormente e - mi rivolgo al collega Gamba - la questione occupazionale

più di qualsiasi altra cosa, se non la salute dei nostri concittadini: a fronte della salute, dobbiamo trovare eventualmente alternative occupazionali che permettano a quella parte del territorio di avere uno sviluppo anche migliore di quello che c'è adesso; mai mettere in contrapposizione occupazione ed ambiente, occupazione e salute. Questo, infatti, è un modo di ragionare antico, oggi non più consono alle indagini e alle ricerche scientifiche, e anche al modo di pensare che finalmente si sta affermando

Presidente, onorevoli colleghi, ricordo a me stesso e agli amici qui presenti che ho l'onore di rappresentare la Sardegna in Parlamento da cinque legislature, e uno dei primi atti che feci da parlamentare fu proprio presentare una mozione sul tema

Rimane il fatto che, ad oggi, non abbiamo ancora la certezza se, per esempio, l'uranio impoverito è stato mai utilizzato nei poligoni

Mi pare che le ultime analisi abbiano dimostrato che l'uranio presente nel territorio non può essere quello che si ritiene impoverito, ma non abbiamo ancora un dato sicuro,

ma anche di salute degli animali. Guarda caso, in quella zona, si riscontrano anomalie alla nascita di animali

anche in altre occasioni) si sta adoperando per ottenere risposte. Rilevo che, per la prima volta, il Governo colloquia con la Regione per fornire risposte. Adesso basta con la demagogia: non utilizziamo il dramma di un territorio per prendere medaglie né nel centrodestra né nel centrosinistra.

Italia dei Valori ritiene si debba andare oltre la verifica della sussistenza di un nesso causale tra particolari fattori patogeni e l'insorgere di gravi patologie nel personale militare e civile procedere piuttosto ad un'opera di bonifica, prevenzione e soprattutto tutela di quanti ormai dalle esposizioni abbiano contratto gravi malattie. Tale ragionamento deve essere fatto anche e soprattutto per la vicenda del poligono di Salto di Quirra, oggetto della mozione in discussione. Tale poligono sorge in un territorio compreso tra le Province di Cagliari ed Ogliastra, nella parte Sud-orientale della Sardegna, e si estende per circa 14.000 ettari. Al suo interno si svolgono da più di 20 anni attività di carattere operativo, logistico e tecnico, oltre che di sperimentazione e messa a punto di velivoli, missili razzi e radiobersagli. Da tempo si è a conoscenza che tali attività, negli anni, hanno prodotto un forte impatto ambientale sul territorio e che, proprio per questo, lo stesso necessita non solo di periodiche attività di bonifica, ma anche di una ferrea e costante attività di controllo, soprattutto alla luce del sistematico utilizzo del poligono da parte di ditte private, fabbricanti d'armi e forze armate straniere che, essendo estranee al territorio e pertanto sprovviste di ogni minima sensibilità o interesse per la tutela e la salvaguardia dello stesso, hanno negli ultimi anni testato armi, munizioni e proiettili all'uranio impoverito, provocando la contaminazione di tutta l'area circostante. Ecco perché il Gruppo dell'Italia dei Valori ritiene necessaria una immediata sospensione delle convenzioni stipulate con tali ditte o forze armate straniere, sospensione che possa portare ad un sereno svolgimento dell'attività della magistratura e ad una rinegoziazione delle medesime convenzioni, prevedendo esplicitamente la revoca di quelle non compatibili con la tutela della salute. La situazione, infatti, è drammatica. Non vi è famiglia che non abbia un parente colpito da linfomi e leucemie. Le indagini condotte sul bestiame attorno al poligono avrebbero rilevato la presenza di agnelli affetti da deformazioni congenite genetiche. Il 65 per cento dei pastori, negli ultimi risulta essersi ammalato di linfoma o leucemia. Oltre ad aumentare il numero dei nati con gravi malformazioni, si contano almeno 21 decessi accertati per tumore tra gli allevatori. Un quadro, come dicevo, terribile che ha indotto il procuratore di Lanusei, Domenico Fiordalisi, ad aprire un fascicolo con ipotesi di reato pesantissime: omicidio plurimo, violazioni ambientali, omissione d'atti d'ufficio in relazione ai controlli sanitari. Lo stesso procuratore ha inoltre disposto, per almeno due mesi, il blocco delle esercitazioni e il sequestro di otto bersagli. Una vicenda, quella del poligono di Salto di Quirra, al centro anche dei lavori della Commissione d'inchiesta sull'uranio impoverito. del Gruppo dell'Italia dei Valori, senatore Caforio, segretario della medesima Commissione, ha provveduto a richiedere l'audizione dello stesso procuratore di Lanusei al fine di incentivare quel percorso di verità e giustizia che riteniamo sia ormai un dovere e una necessità. Noi dell'Italia dei Valori crediamo sia giunto il momento di fare chiarezza sulle omissioni e sulle negligenze che hanno prodotto il silente dramma del poligono di Salto di Quirra. Crediamo altresì che si debbano accertare le responsabilità di chi ha permesso che in quel poligono si facesse e si sperimentasse di tutto dietro pagamento del canone di affitto al Ministero della difesa (1,2 milioni di euro al giorno, come riportato in un *reportage* dal settimanale «Sette» del «Corriere della Sera»). Abbiamo a cuore la salute dei cittadini e chiediamo una maggiore attività di controllo e monitoraggio ambientale nell'area del poligono. Tuttavia, pur votando convintamente a favore della mozione Scanu, alla quale abbiamo appena aggiunto la nostra firma, riteniamo sia doveroso andare oltre la sospensione delle attività missilistiche di sperimentazione e di ogni altra attività addestrativa o operativa, nonché del ripristino di un costante monitoraggio. Crediamo si debba al più presto disporre il sequestro conservativo dell'intero poligono.

Signor Presidente, preliminarmente dichiaro il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico alla mozione di cui è primo firmatario il collega Gamba. Nell'occasione, rinnovo l'apprezzamento e il ringraziamento nei confronti del rappresentante del Governo, non solo per l'importante azione di mediazione

che ha cercato in tutti i modi, riuscendovi peraltro, di fare in modo che ci fosse finalmente in questa fase dei lavori uno stacco rispetto a ciò che è accaduto finora, a ciò che si è verificato inutilmente nelle Commissioni che hanno preceduto quella in attività, per passare dalle parole ai fatti. Io credo che questa non sia una occasione ricca soltanto di celebrazioni e di formalismi. Sono assolutamente convinto del fatto che stasera, con il voto di queste due mozioni, che anche a me piace definire, come ha appena fatto il collega Torri, complementari l'una all'altra, si determinerà l'apertura di una nuova stagione. E ritengo che sia anche una felice condizione, piuttosto che una coincidenza favorevole, il fatto che a rappresentare autorevolmente il Governo in questa circostanza ci sia un sardo, l'onorevole Cossiga. Sappiamo tutti, Presidente e colleghi, quale sia il valore, il significato

che per definizione connotano una mozione, si deve necessariamente unire una passione civile e una tensione ideale, che sono le uniche condizioni a seguito delle quali può nascere la volontà politica. Oggi il Senato si accinge a muovere in maniera consapevole, ragionata ed assolutamente propositiva, all'insegna della ricerca di una comunione effettiva di intenti, un passo importante: il cammino inizia domani. Sono convinto che non solo per il tramite del sottosegretario Cossiga, ma anche per il tramite della Presidenza del Senato e di tutte le forze politiche presenti in questo questo Parlamento, il significato e il contenuto delle mozioni possano inverarsi nella realtà. Facciamo in modo che - perché questo lo dobbiamo e perché lo possiamo

che vivono e lavorano in Sardegna, tutto questo possa finire, tutto questo possa ottenere, per quanto potrà valere,

Signor Presidente, signor Sottosegretario, il Gruppo del PdL mi dà mandato di comunicare che noi voteremo a favore di entrambe

Onorevoli colleghi, è stata convocata la Conferenza dei Capigruppo. In attesa delle comunicazioni della Presidenza, la seduta è sospesa.

Onorevoli colleghi, si è appena conclusa la Conferenza dei Capigruppo che è stata convocata in relazione alla possibile modifica da parte della Camera dei deputati del decreto-legge recante proroga termini, già approvato dal Senato. A tale riguardo, tenuto conto che la data di scadenza del decreto-legge è domenica 27 febbraio, le Commissioni riunite 1a e 5a per la sede referente e la Commissione bilancio per il parere sulla copertura finanziaria sono fin d'ora autorizzate a convocarsi a partire dal pomeriggio di venerdì 25 febbraio. Gli emendamenti all'Assemblea dovranno essere presentati entro le ore 10 di sabato 26. L'Assemblea sarà convocata nella stessa giornata di sabato 26, alle ore 11. Il dibattito, comprensivo di relazioni, discussione generale ed esame degli emendamenti avrà complessivamente la durata di tre ore. Su tale base si procederà alla ripartizione dei tempi. Le dichiarazioni di voto, con trasmissione diretta televisiva, inizieranno alle ore 14, cosicché il voto finale potrà avvenire intorno alle ore 15.